del provvedimento recante "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilita",

riferire sui lavori della Commissione.

vorrei dare alcuni chiarimenti a lei e a tutte le senatrici e i senatori presenti

Sono state poi svolte audizioni, dal 18 febbraio 2020 al 22 luglio 2020,

Al Senato, come il Presidente ricorderà - ma lo voglio ricordare a tutti, perché voglio ricordare i fatti e separarli dalla narrazione che si vuole raccontare al Paese l'assegnazione in sede referente alla Commissione che mi onoro di presiedere è del 5 novembre 2020. Il primo sollecito, la prima richiesta di calendarizzazione di questo testo risale al 13 gennaio 2021, un po' di mesi dopo. Qualcuno dirà che non si poteva fare prima, perché c'era la sessione di bilancio. Va bene, ricordo che qualcuno accusa di aver rallentato i lavori, perché nell'aprile di quest'anno, il 2021, è avvenuto un fatto - sempre un fatto, non una narrazione c'è stata una lettera, inviata da me, su incarico di tutto l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al Presidente del Senato, nella quale si dava atto della presenza di ulteriori disegni di legge, che vertevano sulla stessa materia, che dovevano essere congiunti al testo in esame, il disegno di legge Zan, che arrivava dalla Camera siccome erano in sedi diverse, per essere congiunti dovevano prima essere riassegnati. Questo non lo dice il presidente Ostellari, ma lo dice il Regolamento del Senato, all'articolo 51.

ci sono i documenti: la programmazione dei lavori parla chiaro, essa viene inviata a tutti i Capigruppo della Commissione. Quel problema, se lo si voleva risolvere, lo si poteva risolvere prima. Ma tant'è. Andiamo avanti; siamo quindi al 7 aprile 2021. La risposta del Presidente arriva il 13 aprile 2021; subito dopo la sua risposta, signor Presidente, noi non abbiamo tardato. Infatti il 27 aprile, con l'ufficio di programmazione dei lavori, che ho dovuto fare perché ovviamente di programmazione integrato dai Capigruppo non c'era l'unanimità, ho dovuto far votare in Commissione plenaria il calendario dei lavori, cosa che di solito non si fa. fa. Per problemi legati ovviamente a diverse opinioni sul calendario e sull'opportunità del calendario stesso, ho dovuto procedere così, come da Regolamento. Il 28 aprile questo testo è stato messo nel calendario della Commissione e da lì si inizia a lavorare in Commissione sul testo. Sono state fatte richieste di disgiunzione dei testi e richieste di congiunzione del nuovo testo a firma Ronzulli. Ebbene, nel mese di maggio sedute dedicate a questo provvedimento, mentre nel mese successivo sono state dedicate alle audizioni ben sette sedute, con 60 persone audite.

di costituzionalisti e di educatori; abbiamo potuto ascoltare persone che non erano state sentite alla Camera, perché vi ricordo che questo provvedimento non è quello che è stato oggetto di audizione alla Camera dei deputati. Questo provvedimento è uscito dalla Camera dei deputati e oggi ce lo troviamo qui. Attraverso queste audizioni abbiamo potuto comprendere, signor ci sono dei motivi ideologici. Io non sono chiamato a esprimere oggi un giudizio su questo; lo farete voi, lo faremo dopo nella discussione. Ci sono degli evidenti problemi di ordine tecnico-giuridico, che sono emersi tutti nella medesima direzione: dalle associazioni di femministe, Arcilesbica, costituzionalisti, professori, educatori.

Essi si concentrano, signor Presidente, su tre punti fondamentali: l'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 7. In questo modo noi, attraverso le audizioni, abbiamo aperto il dibattito. Evidentemente forse non era possibile farlo prima, perché c'erano quei problemi regolamentari. Ma l'abbiamo potuto fare oggi e registrare oggi, in questi giorni, grazie a questo lavoro. Cosa accade poi? È arrivata anche una nota verbale dalla Santa Sede, che è stata acquisita al nostro fascicolo e che le ho consegnato per conoscenza, signor

E pur di trovare una soluzione, signor Presidente, a quel punto abbiamo fatto anche un tavolo politico. E il tavolo politico, formato ovviamente dalle forze di maggioranza che sostengono questo Governo, ha fatto emergere, intanto, la disponibilità:

Forza Italia e Italia Viva. A seguito di queste osservazioni, quindi, ho potuto lavorare su una ipotesi di mediazione che, ovviamente, teneva conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi Gruppi e di ciò che abbiamo sentito dalle audizioni. Ho, quindi, depositato, in quel contesto, una proposta di mediazione; una proposta che, come lei ricorderà e come ricorderanno tutti, ha ricevuto una

è stato anche suggerito, da parte della senatrice De Petris, nonostante il calendario fissato per oggi e votato allora, di procedere al deposito della proposta che avevo presentato presentato in quel tavolo politico. Io, allora, sono andato in Commissione, ho colto l'invito della senatrice De Petris e ho illustrato quella che era la proposta. Quindi,

come testo base e su quello si operano sostanzialmente tre modifiche. Qualcuno le ritiene troppo invasive, qualcun altro meno, ma quella è la strada. Quella è la strada, dettata da costituzionalisti, da professori, da associazioni, da educatori e anche dalla Santa Sede. Certo che siamo uno Stato laico, ma questo non è in discussione. Non è questo il tema. Il tema è verificare se quei problemi di ordine giuridico sono problemi che intendiamo risolvere oppure no. Signor Presidente, la

Questa disponibilità politica, a mio avviso, nella maggioranza esiste. C'è qualcuno che, evidentemente, forse mira a impedire l'approvazione di un buon testo. Io dico che, a fronte del lavoro che abbiamo fatto, oggi è mio dovere rappresentare all'Aula questa necessità di provare fino all'ultimo la volontà politica di dialogo.

se c'è la disponibilità a continuare quel dialogo che avevamo intrapreso in quel tavolo politico che aveva dato ottimi frutti, sulla base del quale in brevissimo tempo, secondo me

sollevate da molti e forse da troppi

nella Commissione giustizia sul disegno di legge Zan. Alla luce di quanto lei ha affermato, per capire qual è la volontà politica dell'Assemblea, sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza

di un provvedimento importante che riguarda diritti umani e diritti civili, non altro; serve a proteggere (solo a questo serve) a questo serve) delle persone deboli per la propria condizione e per la propria natura, che spesso vengono discriminate e subiscono violenze. Non è quindi opportuno, Presidente, che su questo si facciano giochini politici o strategie. Io mi sento in dovere di raccontare all'Assemblea cosa è successo, aver letto i giornali in questi otto mesi per sapere cosa è accaduto in Commissione. Ci è stato impedito di discutere fino a marzo

Ci è stato detto che quel disegno di legge non doveva andare avanti perché era divisivo nella maggioranza, poi si è cercato di congiungerlo, poi sono state fatte 170 audizioni - ha ragione Ostellari - tutte uguali.

un provvedimento che riguarda la vita delle persone *(Applausi)* e i giochini, le tattiche e le furbizie vanno chiusi. Adesso basta, Presidente, si è deciso un percorso, lo si faccia in Assemblea e lo si faccia bene. Purtroppo in Commissione non ci sono state le condizioni neanche per aprire la discussione.

finestra"). Colleghi, vi inviterei a tenere la calma. C'è già un clima incandescente. Io do la parola a chi mi chiede di parlare. Visto che c'è stato un intervento piuttosto lungo e dettagliato, qualcuno ha contrapposto qualche altra cosa; io poi decido quello che voglio fare. Rispettiamo l'ordine delle richieste.

Presidente, dobbiamo ristabilire la verità in Assemblea perché non è possibile...

Presidente della Commissione di dare la sua versione, doveva dire qual è lo stato dei lavori, non può egli fare la storia, tra l'altro non corretta, di tutti quelli che sono stati i lavori in Commissione. in Commissione dal centrodestra che non si doveva nemmeno trattare un provvedimento che era stato votato dalla Camera. *(Applausi)*. Abbiamo dovuto forzare e chiedere voti

di non essere esasperati, ma all'esasperazione porta il comportamento di un Presidente di Commissione che più volte ha calpestato le prerogative della Commissione stessa *(Applausi)* quando quando ci ha impedito la stessa calendarizzazione del provvedimento in discussione.

Presidente, al di là del balletto dei numeri - quattro mesi, otto mesi, un anno, non importa agli atti c'è una Commissione giustizia che è stata calpestata nelle sue prerogative. *(Applausi)*. Il Presidente ci ha impedito persino la votazione sulla calendarizzazione. Ora noi a grandissima fatica abbiamo votato. L'Assemblea si è espressa

Aggiungo che la mediazione sarebbe possibile se chi vuole mediare fosse davvero interessato a tutelare i diritti delle persone in questione, ma così non è.

*(M5S)*. I maggiori esponenti del partito della Lega hanno sempre negato pubblicamente che il problema dell'omotransfobia esista, per cui il loro interesse oggi sulla questione è assolutamente incredibile. *(Applausi)*. Presidente, Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia è molto sereno. Non ha partecipato a questa parte molto nervosa dei Ha preso atto della sua cortesia nei confronti del collega del PD che ha chiesto di intervenire quando lei aveva già sospeso la seduta.

non abbiamo interrotto nessuno. *(Proteste)*. Il Gruppo Fratelli d'Italia non ha minimamente partecipato alla prima fase nervosa

- viene accusato dai componenti stessi della Commissione di non so quali misfatti - si lamenta - e questo è un dato storico - del fatto che l'esame di merito è stato sospeso con un voto del Senato per portare in Aula un provvedimento che era ancora all'esame della Commissione. Quindi, semmai, dovrebbe lamentarsi chi non ha potuto svolgere appieno - secondo alcuni in maniera troppo lenta

Conferenza dei Capigruppo per verificare la legittima richiesta di un Presidente di Commissione...

sono d'accordo - provvedimento, nel quale per alcuni si discute delle fragilità e per altri anche del diritto di opinione *(Applausi)*, della possibilità di esprimere le proprie idee: questo è un dato di fatto. è un dato di fatto. Per alcuni c'è la mascherina col tricolore e per altri solo quella con i colori dell'arcobaleno *(Applausi)*, come voi dei 5 Stelle: questa è la verità. signor Presidente, la prego di riconfermare la sua decisione, che per noi è indifferente, perché - lo ricordo - abbiamo accettato la valutazione e abbiamo presentato una pregiudiziale di incostituzionalità

proprio per capire lo stato dell'arte del disegno di legge Zan. Ma poiché è stata convocata alla stessa ora la Commissione giustizia, ho detto che l'avrei rinviata. Quindi, la polemica di oggi è assolutamente pretestuosa, perché era già stata annunciata la mia volontà nella *chat* comune dei Capigruppo. Questo lo dico per chiarezza: la mia decisione è già presa. Presidente, personalmente mi autocensuro perché ritengo che tutti gli interventi sull'ordine dei lavori non lo fossero e non avrebbero dovuto esserci, perché lei ha disposto la convocazione della Capigruppo e la sospensione della seduta e, quindi, *tamquam non esset* rispetto a quello che è accaduto.

all'interno di una stanza dove non ci sono telecamere e non si registra quanto diciamo, può veramente essere esperito il tentativo della ricerca di una mediazione. Non sarà una cosa evidente, forse non ci saranno bandierine. Ma, se qualcuno vuole raggiungere un risultato serio e concreto sull'argomento, quella è la sede propria della politica dove trovare una soluzione.

di poter interloquire con i colleghi, con una modalità - direi - un po' informale ma importante, per chiarire alcuni punti prima di riunirci tra noi Capigruppo. È assolutamente vero, signora Presidente, che lei ce lo aveva già anticipato: ci aveva anticipato che ci saremmo riuniti e devo dire che la richiesta del presidente Ostellari... *(Brusio).* Vi chiedo scusa, colleghi: vi chiedo solamente pochi secondi del vostro tempo, consapevole del fatto che siamo formalmente in sospensione dei lavori, solamente per precisare, a nome del Gruppo che rappresento, alcuni punti secondo me utili per il prosieguo della discussione in Capigruppo e anche in Aula. Condivido la richiesta del presidente Ostellari, perché ancora una volta la settimana scorsa, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, abbiamo avanzato esattamente la seguente proposta: abbiamo chiesto che si partisse, già dalla settimana scorsa, per una mediazione su di un testo solo parzialmente condiviso, ma come buona base di partenza. *(Commenti)*. Collega De Petris, chiedo scusa se mi rivolgo direttamente a lei, ma hanno parlato tutti: chi si chiama democratico deve agire di conseguenza. Un po' di cortesia. già dalla settimana scorsa avremmo potuto cominciare a lavorare su questo testo e avremmo già una settimana di vantaggio su quella mediazione che va non nel nostro interesse, ma nell'interesse di quelle persone, i destinatari della norma, della norma, che voi dite di voler tutelare. Colleghi, prima di riunirci in Capigruppo, vorrei precisare due cose: in primo luogo, nessuno in quest'Aula ha il diritto di dare patenti di tutela dei diritti fondamentali più o meno buona, più o meno efficace, più o meno lecita, ad alcuno. *(Applausi)*. Se vogliamo essere precisi - e me ne scuso - sicuramente non quella parte che la scorsa legislatura non ha votato le unioni civili, a differenza di chi parla. *(Applausi)*. Quindi, cortesemente, nessuno si permetta di fare delle considerazioni, di dare delle patenti o di fare analisi del sangue che sono assolutamente fuori contesto in questa fase. Noi non ci stiamo Seconda considerazione: se veramente vogliamo fare una mediazione - e noi lo vogliamo, perché non riteniamo che questa discussione debba limitarsi alla porzione di mondo buona che rappresentate voi e la porzione di mondo cattiva che rappresentiamo noi - perché vogliamo dare alla norma un aspetto più compatibile con la sua efficacia, chiediamo ancora una volta che la norma venga discussa in quest'Aula e non solo in maniera apparente, formale e senza modifiche, mantenuta in un testo che noi riteniamo non solo inutile, ma pericoloso proprio per i suoi destinatari, proprio per quella libertà di espressione di cui tante volte si è parlato in quest'Aula e che a volte così poco si rispetta. Non esiste un'unica verità, colleghi: lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Non esiste un'unica ragione, la vostra. Esistono le libertà, i diritti, le opinioni anche di chi la pensa diversamente da voi. E questo elemento di democraticità fondamentale deve emergere anche da questa norma che noi reputiamo importantissima come atto di civiltà giuridica. Al presidente Grasso dico che davvero non siamo riusciti a sentirlo, ma è stato un elemento acustico, non politico. Purtroppo non siamo riusciti ad ascoltare il suo intervento e ci dispiace, anche perché è molto atipico che tutto questo avvenga non in una fase di discussione generale, ma in una fase in cui la seduta avrebbe dovuto essere sospesa. È evidente che, se parla la parte che si arroga il diritto di essere la migliore e l'unica depositaria della verità, anche noi dobbiamo dire la nostra e spiegare perché fino alla fine, proprio per difendere i diritti dei destinatari di questa norma che a noi stanno a cuore, continueremo a lottare per una vera mediazione, che è non ostruzionismo, ma vera tutela dei diritti.

Come vogliamo educare le persone con la Giornata contro la discriminazione e contro l'odio se non siamo in grado di risolvere la questione e parlarci civilmente per ottenere una soluzione?

con tutto quello che abbiamo da fare, dalla procedura civile ai decreti che scadono. Mi chiedo se vogliamo veramente continuare in questo clima, oppure fare tutti un piccolo passo indietro e magari rinunciare a una parola,

autore di queste discriminazioni e invece stiamo discutendo di tutt'altro. Mi sembra un incontro di *wrestling* a favore di telecamere con finte botte. Credo che invece abbiamo il dovere - come lei ci ha chiesto, Presidente, in Conferenza dei Capigruppo - di verificare se c'è un percorso positivo da poter fare insieme per dotare il Paese di una legge che tuteli persone che soffrono soltanto perché vogliono esprimere liberamente il proprio amore. Questo è il tema. Per il resto, forze politiche che pensano di poter

fino a mercoledì 21 luglio. Il prosieguo della seduta odierna prevede la discussione di questioni incidentali presentate sul disegno di legge sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità, fino alle ore 20. L'esame del provvedimento proseguirà domani, a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 20, e giovedì 15 luglio, dalle ore 9,30. La seduta di giovedì si concluderà con il *question* *time,* che prevede la presenza dei Ministri dell'istruzione, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale. Gli emendamenti al disegno di legge n. 2005 dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 20 luglio. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre, alle ore 16,30, la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 19,30. Il calendario della prossima settimana prevede, nella giornata di martedì 20 luglio, dalle ore 16,30 fino alle ore 20, il seguito della discussione generale del disegno di legge n. 2005. Nella giornata di mercoledì 21 sarà discusso il decreto-legge imprese, lavoro, giovani e salute, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati. In base alle ultime disposizioni adottate dei senatori Questori,

l'articolo 1 del disegno di legge Zan viola l'articolo 3 della Costituzione e questo non lo dico io, lo ha detto, durante le audizioni, un insigne giurista del calibro di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. La nostra Costituzione, cari colleghi, parla di tutela della persona in base al sesso che è una condizione oggettiva. di legge Zan troviamo scritto che accanto al sesso - che intanto non è più il sesso biologico come tutti noi siamo abituati a ritenere, ma automaticamente può essere biologico o anagrafico, e già qui

orientamento sessuale e identità di genere. Queste definizioni non sono giuridiche, non hanno una qualità giuridicamente riconoscibile, sono definizioni date sulla base di teorie filosofiche o

detto nel disegno di legge Zan all'articolo 1, dove si legge che: «per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Questa norma, di fatto, permetterà a chiunque di autopercepirsi sulla base della convenienza del momento, violando evidentemente qualsiasi criterio di oggettività nella propria definizione. Questo non è l'unico problema di costituzionalità di questa norma. Ve ne sono molti altri. L'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini la libertà di pensiero, la libertà di parola e la libertà di espressione. gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge Zan fanno esplicito riferimento alla modifica degli articoli del codice penale introdotti con la legge Mancino-Reale. Peccato, cari colleghi, che la legge Reale-Mancino faccia riferimento a caratteristiche della persona oggettivamente riconosciute come, ad esempio, la razza, la religione o l'etnia. Non possono essere riferite a una legge gravemente punitiva come la legge Mancino-Reale caratteristiche che, come detto, sono di sostanziale autopercezione della persona. Io, però, Presidente, mi permetto di chiedere, se possibile, che davanti a un tema così importante, così dibattuto e per il quale il Paese si è spaccato a metà l'Assemblea abbia la gentilezza di ascoltare, che i colleghi abbiano la gentilezza di ascoltare, visto che oltretutto il dibattito in Commissione è stato brutalmente fermato. Quindi che almeno in Aula ci si ascolti, se possibile,

ai colleghi che sostengono questa proposta di legge se sarà ancora possibile parlare, per esempio, di contrarietà al matrimonio tra persone dello stesso sesso, se sarà ancora possibile esprimersi pubblicamente contro l'adozione da parte di coppie *same sex*, oppure se sarà ancora possibile dichiararsi contrari alla maternità surrogata, *alias* utero in affitto, utero in affitto, oppure se tutto questo sarà letto come istigazione alla discriminazione, perché la fattispecie di istigazione alla discriminazione è talmente fumosa, talmente difficile da definire in modo tassativo che tutto potrà essere considerato istigazione alla discriminazione, anche perché, come abbiamo sentito proprio nel dibattito di questi giorni, qualcuno sta già dicendo che i diritti riproduttivi sono diritti inalienabili della persona. Conseguentemente, dirsi contrari all'adozione da parte di coppie *same sex* o dirsi contrari alla maternità surrogata diventerà evidentemente un'istigazione alla discriminazione; sarebbe come se qualcuno venisse a dirmi che io non mi devo riprodurre: sarebbe sì istigazione alla discriminazione. Peccato che in questo caso l'attenzione del legislatore non deve essere verso i diritti della coppia *same sex*,

ha diritto a non essere acquistato su Internet. Ancora. Alcune critiche, a mio avviso sensate e assolutamente condivisibili, sono venute da illustri costituzionalisti anche con riguardo all'articolo 4 di questo disegno di legge:

ma nella seconda parte si va a limitare il dettato costituzionale dicendo che quelle opinioni non possono essere idonee a determinare il concreto pericolo di atti discriminatori. il senatore Pillon che, come ben sapete, è dipinto da tutti i giornali come pericoloso omofobo, ma lo dice un giurista del calibro del presidente emerito della Consulta Mirabelli - si tratta di una limitazione del dettato costituzionale inaccettabile. Inoltre, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge Zan vanno anche contro il dettato costituzionale dell'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce la tassatività della norma penale. Mi permetto di aggiungere una considerazione a quanto troverete scritto nella nostra questione pregiudiziale di costituzionalità: siamo sicuri che usare lo strumento penale anche in questo caso sia la strada giusta? Vedete, abbiamo forse preso una brutta abitudine, che è quella di usare sempre e solo lo strumento penale come se fosse il miglior modo per educare il popolo.

Ci sono parole, come quelle che abbiamo ascoltato dal presentatore del disegno di legge Zan, che leggo testualmente: ci sono dei bambini che percepiscono il proprio genere, fin da quando sono bambini, diversi dal loro sesso; ecco che allora bisogna aiutare i bambini in un loro percorso di transizione. Sono parole che ci

associazioni di militanti lesbiche e associazioni di militanti femministe hanno fatto pervenire alla nostra Commissione; preoccupazioni che avremmo voluto poter ascoltare e poter valutare per arrivare a un testo che fosse accettabile; preoccupazioni che non avete voluto ascoltare e che ci inducono a dire che questo disegno di legge va fermato perché così non va. ha detto il presidente Draghi - controlli preventivi nelle Commissioni parlamentari che garantiscono circa il rischio di violazione dei trattati. Bene, attiviamo quei controlli preventivi, perché non sono stati attivati.

perché siamo veramente preoccupati di alcuni passaggi di questo disegno di legge che a nostro giudizio violano palesemente alcuni articoli fondamentali della Costituzione. In particolare, l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce il diritto di pensiero e di manifestazione delle proprie opinioni viene, a nostro avviso, messo in pericolo dall'articolo 2 del disegno di legge, il quale non punisce - badate bene - la violenza e l'istigazione alla violenza nei confronti di una persona soltanto in ragione del suo orientamento sessuale, ma punisce anche l'istigazione alla discriminazione, l'istigazione alla discriminazione, senza che in questo disegno di legge sia in alcun modo spiegato in cosa esattamente consista. Se noi leggiamo l'articolo 2 disegno di legge comprendiamo l'assoluta indeterminatezza di questa norma, perché l'articolo 1 definisce l'orientamento di genere come una autopercezione e una autodichiarazione assolutamente soggettiva e slegata da qualsiasi parametro biologico od oggettivo. Allora voi capite bene, colleghi, che il combinato disposto di queste due norme comporta una norma penale in bianco, che potrà essere riempita discrezionalmente da qualsiasi magistrato a seconda del suo orientamento, dei suoi convincimenti, delle sue posizioni morali, religiose, etiche, politiche o filosofiche. Stiamo cioè confezionando una norma per imbavagliare chiunque la pensi diversamente dal magistrato che di volta in volta giudicherà su quel caso. Questo è il vero rischio che oggi stiamo mettendo in atto qualora dovessimo approvare questa norma. norma. Fratelli d'Italia - ripeto - è pronta a votare anche oggi una norma che aggravi, anche pesantemente, le sanzioni nei confronti di chi commette violenza o istiga alla violenza, ma non è assolutamente disposto a votare una norma che creerà inevitabilmente un reato di opinione, violando l'articolo 21 della Costituzione. Costituzione. Cari colleghi, di questo siete consapevoli anche voi, sostenitori di questo disegno di legge, perché altrimenti non avreste sentito il bisogno di scrivere l'articolo 4, l'articolo 4, che non fa altro che sancire - in modo più confuso peraltro - quello che sancisce l'articolo 21 della Costituzione. Che bisogno c'è di richiamare l'articolo 21 della Costituzione all'interno dell'articolo 4 del disegno di legge, dato che anche i bambini sanno che la Costituzione prevale sempre su ogni legge, essendo una fonte del diritto sovraordinata? Che bisogno ci sarebbe di inserire l'articolo 21 della Costituzione dentro l'articolo 4 del disegno di legge, se gli stessi sostenitori di questo provvedimento non si rendessero conto del rischio che comporta questa norma nel reprimere legittime opinioni in ordine di famiglia naturale, in ordine del diritto di un bambino di avere un padre e una madre, in ordine di gestazione per altri o utero in affitto che dir si voglia, in ordine al fatto che lo Stato deve sostenere soltanto la famiglia naturale? Fermo rimanendo il diritto di chiunque di fare ciò che crede nella propria vita privata, la funzione sociale della famiglia fondata da un uomo e da una donna per mantenere, istruire, educare e allevare un figlio è un'altra cosa. *(Applausi)*. E noi vogliamo avere il diritto di continuare ad affermare questi nostri convincimenti senza che qualcuno ci metta sotto processo.

di discriminazione o di violenza. Ma chi stabilisce se esiste o meno questo rischio, questo pericolo? Ovviamente lo può stabilire solo un magistrato, signor Presidente. Questo vuol dire che chiunque di noi dica, ad esempio, che un bambino ha diritto ad avere una madre e un padre potrebbe domani trovarsi denunciato da una associazione di omosessuali, di *gay* o altro che si sente discriminata da questa nostra affermazione e il magistrato lo dovrà rinviare a giudizio e lo dovrà giudicare. Cosa dovrà giudicare, cari colleghi? Dovrà giudicare un fatto, sulla base del principio di tassatività dell'articolo 25, secondo comma della nostra Costituzione o dovrà giudicare un'opinione,

filosofico o se l'abbia fatto animato da motivi di odio? Questo dovrà giudicare il magistrato. State creando una norma per giudicare lo stato d'animo interiore dell'imputato. Negli ordinamenti giuridici conosciuti nel mondo intero questo istituto si chiama diritto penale dello stato d'animo interiore è stato applicato in due soli ordinamenti, cari colleghi: nell'ordinamento giuridico nazionalsocialista e nell'ordinamento giuridico della Russia sovietica, che poi ovviamente ha ispirato tutti gli altri regimi comunisti del mondo. Solo in questi due ordinamenti giuridici non si giudica un fatto, ma si giudica uno stato d'animo. Noi dovremo andare a giustificare davanti a un giudice il nostro stato d'animo. Questo è quello che voi state introducendo con questo disegno di legge. Certo, speriamo e confidiamo di trovare un giudice ragionevole, un giudice che magari non antepone le sue convinzioni

sotto processo del tutto ingiustamente. Il risultato di tutto questo sarà quello a cui, in realtà, vuole mirare la maggioranza: l'autocensura. Quando gli italiani sapranno che parlare di certi argomenti comporta il rischio di un processo penale si autocensureranno, non si avventurano più su un terreno minato e quindi il politicamente corretto trionferà,

di diritti dei minori la pensa esattamente come noi, ma il politicamente corretto chiuderà loro la bocca, come ha certificato anche un recente sondaggio negli Stati Uniti, dove due elettori repubblicani su tre hanno dichiarato di non parlare più di questi argomenti in pubblico per paura della reazione che verrà inevitabilmente manifestata nei loro confronti. Con il risultato che avremo una dittatura della minoranza sulla maggioranza. *(Applausi)*. Cari colleghi, questo state preparando con questo...

temi che ci preoccupano molto; ce ne sono anche altri e, in particolare, l'articolo 7, che rischia di aprire le porte delle scuole di ogni ordine e grado alla propaganda *gender*; rischia di mettere i nostri bambini - ai quali non insegniamo l'educazione sessuale perché con questa legge vogliamo insegnare loro l'educazione *gender* - nelle mani di associazioni che probabilmente non sono le più qualificate

membri del Governo, onorevoli colleghi, Italia Viva voterà contro la questione pregiudiziale e con questo potrei cavarmela. Ci sono, però, dei momenti nella vita delle istituzioni democratiche in cui dobbiamo ricordarci chi siamo. Noi non siamo degli *influencer* che mettono i *like*; non siamo delle persone che pensano che la politica faccia schifo

Cerchiamo di essere chiari fino in fondo guardandosi negli occhi e ricordandosi con che faccia siamo andati di fronte agli elettori. Noi abbiamo promesso e giurato sulla Costituzione di servire questo Paese con disciplina e onore. Alla luce di questo, in determinati momenti della nostra vita abbiamo fatto delle scelte che sono state dei compromessi rispetto anche alle nostre idee. Io sono senatore come voi; nella scorsa legislatura non lo ero. Da Presidente del Consiglio dei ministri, il 27° della storia repubblicana, ho posto la questione di fiducia perché si potesse arrivare all'approvazione della legge sulle unioni civili, che io, cattolico, ho firmato,

il provvedimento e che poi, all'improvviso, per qualche telefonata di qualche alto prelato, cambiò posizione. *(Applausi)*. Non prendo lezioni da chi allora cambiò opposizione, perché la storia non si cancella,

però non ho perso il gusto di guardarmi allo specchio. Ora, siamo in un punto delicato; prima di ragionare del provvedimento - siamo in fase di pregiudiziale - dico questo: da otto anni è in discussione una legge che colpisce i reati di omotransfobia, e questa legge è stata approvata dalla Camera dei deputati nel 2013 (primo firmatario Ivan Scalfarotto); quella legge al Senato non ha trovato i voti. Oggi siamo nel 2021: quanti ragazzi omosessuali, transessuali, persone con disabilità - lo voglio dire, perché grazie a Lisa Noja e al lavoro della Camera c'è anche la previsione sulla disabilità - quanti in questi otto anni non hanno avuto quella tutela perché sono mancati i voti? Ve lo dico io: tante e tanti. Oggi siamo nella stessa condizione; siamo a un passo, a un centimetro. Qui non ragiono delle mie idee; ragiono di un'altra cosa: ragiono di politica. Forse fate di quest'Aula un luogo dove gli ultras si confrontano e non si porta a casa il risultato?

o si va a scrutinio segreto - ed è un rischio per tutti - o ci si assume la responsabilità politica di trovare un accordo. L'accordo non è semplicemente nel merito, che è a portata di mano, perché non dobbiamo prenderci in giro: l'accordo è a portata di mano, è a un passo dal traguardo. Il punto non è soltanto l'accordo di merito; è anche un accordo di metodo. Va chiesto a tutte le forze parlamentari non solo di venirsi reciprocamente incontro, ma di fare un patto politico perché alla Camera questa legge, ove venisse modificata dal Senato, possa essere approvata nel giro di due settimane. Colleghi, sono in una fase della mia vita in cui non ho più problemi di ricerca di popolarità, e si vede; sono in una fase della mia vita in cui non ho paura di dire le cose senza ipocrisia. A me quei ragazzi stanno a cuore. Quelle persone, donne e uomini, che rischiano di non avere tutela, oggi sono nelle nostre mani. Se volete piantare una bandierina ideologica perché ve l'ha chiesto qualcuno, ditelo, ma è un'altra storia rispetto alla nostra. Se volete fare ostruzionismo, ditelo, ma non ci prendete in giro facendoci perdere tempo. Se vogliamo trovare un punto di sintesi, io vi richiamo e mi richiamo, signor Presidente, all'alta responsabilità che abbiamo,

è un appello molto semplice *(Commenti)*: si faccia un accordo sui punti legati agli articoli 1, 4 e 7, e, fatto l'accordo sugli articoli 1, 4 e 7, si chieda a tutte le forze politiche di portare la discussione alla Camera entro quindici giorni. Se facciamo questo, avremo dimostrato che la politica non fa schifo. Se si andrà allo scontro, al muro contro muro, e si perderà a scrutinio segreto, avrete distrutto le vite di quei ragazzi.

Avremmo voluto che questo spazio ci fosse anche in Commissione. Il presidente Renzi adesso ha giustamente ricordato che c'è il bicameralismo, per cui chiedere al Senato - e un domani in un'altra occasione potrebbe essere la Camera - di

dobbiamo approvare ciò che pensiamo sia giusto e non approvare ciò che pensiamo sia sbagliato, oltre a cambiare ciò che pensiamo sia modificabile. Tuttavia, la discussione e le questioni si sono evolute in un modo che noi non approviamo veramente in nessun modo. c'è il bicameralismo, il bicameralismo comprende anche le Commissioni. La Costituzione dice che ogni provvedimento va discusso Nelle Commissioni non siamo potuti neppure arrivare agli emendamenti; è vero, abbiamo fatto numerose audizioni,

ma tra i massimi dirigenti ed esponenti del Partito Democratico. Ebbene, questo provvedimento è rimasto lì. Non usate dunque questi scandali, questi problemi procedurali a sproposito. Volete questo provvedimento per ragioni che io davvero non riesco a capire; lo volete immutato e immutabile, come se fosse un testo sacro, anche di fronte a proposte di grandissima apertura. La proposta del presidente Ostellari, ad esempio, era quella di togliere le parole «identità di genere». No, l'identità di genere è intoccabile: senza questo riferimento verrebbero escluse 400.000 persone.

Direi che si allarga un po' il campo e bisognerà fare allora un piano per le prigioni estremamente ampio; se tutti gli omofobi e transfobici, incluso l'onorevole Zan, vi dovranno andare dentro, direi che forse dovremo attrezzare delle piccole aree del Paese per quelli che stanno fuori dalle prigioni.

Pertanto, noi che auspichiamo una soluzione positiva ed equilibrata, di fronte a questo modo di portare avanti la questione siamo davvero molto delusi e vediamo che non è possibile fare un lavoro positivo. Ci troviamo anche in una condizione per cui c'è un accanimento su ogni singola iniziativa portata avanti dal centrodestra. È stato addirittura attaccato il presidente Ostellari, che non avrà fatto probabilmente tutto ciò che alcuni

nessuno! Non è stato detto, ma sono state fatte accuse generiche di menare il can per l'aia, perché forse sarebbe stato parziale. Sappiamo però benissimo che tutti i Presidenti di Commissione appartengono e sono espressione di forze politiche. Colleghi, forse il problema per voi è che la pensi in modo diverso: che poi faccia il Presidente in modo inoppugnabile, per voi non è un problema.

di animosità, a dire poco, nell'esame di un provvedimento che dovrebbe promuovere la tolleranza e l'accettazione del diverso. Il diverso non è soltanto l'omosessuale o il transessuale, ma anche chi la pensa diversamente che ha diritto a non essere insultato, anche se porta avanti posizione diverse. Devono essere rispettati i diritti delle famiglie, devono essere ascoltate le associazioni familiari e tutti coloro che sono espressione della nostra società e non solo certe associazioni di un certo tipo, scelte accuratamente. Non si tratta soltanto delle associazioni LGBT, perché tra queste c'è anche Arcilesbica, che però è stata cassata, non è stata sentita, non è stata ascoltata e non si è dato minimamente retta a quanto ha chiesto. Ecco perché voteremo

ad articoli costituzionali, a norme italiane ed internazionali e alle libertà. Vorrei quindi parlare ai colleghi senatori e alle colleghe senatrici, per due minuti - non per venti minuti chiedendo di superare gli steccati ideologici e guardandoci in faccia. Io non penso che in quest'Aula ci sia un solo senatore, al di là dei partiti, che discrimini in base al sesso. E, se c'è qualcuno che discrimina un essere umano in base al sesso e alla sua scelta di vita, è un cretino che non merita di stare dentro quest'Aula. Noi, come Lega, abbiamo in carica stasera, a metà luglio, parlamentari, sindaci e governatori omosessuali; ne avremo altri. Quando io, da segretario della Lega, firmo le liste, non chiedo: «Sei omosessuale? Sei eterosessuale? Come ti percepisci?». Io cerco di trovare donne e uomini in gamba, senza ghettizzare alcuno, senza etichettare alcuno. *(Applausi)*. E davvero, quando leggo le testimonianze di ragazzi e ragazze

Stavo dicendo che io, come voi, ringrazio i promotori di questa legge e spero che il tratto finale di questo percorso ci veda insieme, perché sarebbe un bellissimo segnale. Che questa sera ci siano ragazze e ragazzi che hanno paura di dichiarare al mondo come vivono il loro amore è drammatico. A me dei giocatori che hanno vinto la finale degli europei domenica sera frega men che zero che gusti sessuali abbiano, e non lo vado a chiedere a Donnarumma, a Chiellini o a Bonucci. Ed è drammatico che in alcuni settori del nostro lavoro e della nostra vita, nell'Italia evoluta e moderna del 2021, ci sia qualcuno, uomo o donna, che abbia paura a dichiararsi *gay* o lesbica perché qualche coglione è pronto a discriminare, ad accusare, a indicare, ad additare,

il diritto alla libertà con la L maiuscola, poniamo un attimo da parte la bandiera, l'ideologia e il paraocchi.

Se ci sono stasera a passeggio per le strade di Roma due ragazzi che si baciano o due ragazze che si amano e si prendono per mano, nessuno si può e si deve permettere di ironizzare, di offendere e men che meno di aggredire quei ragazzi e quelle ragazze. *(Applausi)*. Vogliamo aumentare le pene per queste persone? Sì, assolutamente. Io ho due figli: come cresceranno i miei due figli e chi ameranno i miei due figli è affare loro. Io mi sono preoccupato, nei limiti del possibile, da genitore separato e divorziato, di dare loro i fondamenti del rispetto e della buona educazione. Il lavoro che faranno e la donna o l'uomo che ameranno saranno affar loro. E saranno miei figli, e le loro compagne e i loro compagni saranno in casa mia come in casa loro. *(Applausi)*. Se siamo d'accordo su questo, smettiamola. Prendiamocela piuttosto con quei Paesi al mondo - e purtroppo ce ne sono ancora troppi - che per l'omosessualità prevedono la pena di morte, l'ergastolo o il carcere. Ridiscutiamo gli accordi commerciali con quei Paesi. Io non voglio fare affari con l'Iran, dove l'omosessualità è punita con la pena di morte. No, mi rifiuto.

prendiamo la parte più importante, per la quale ringrazio il collega Zan. Togliamo quello che divide non solo quest'Aula, ma tutto il Paese. Togliamo i bambini togliamo l'educazione affidata alle scuole elementari: lasciamo alla mamma e al papà il diritto e il dovere di educare i propri bambini, non allo Stato. Decideranno loro, da grandi, cosa fare, come amare e chi amare. Togliamo i bambini, togliamo le scuole elementari e togliamo un reato. Tra l'altro, se qualcuno in quest'Aula si sente al di sopra della legge, perché tanto a lui non capiterà mai non vorrei portare sfortuna - dico che noi dobbiamo approvare delle leggi oggettive. Meno spazio di interpretazione lasciamo ai giudici e ai tribunali, meglio è. Un reato deve essere chiaro.

per la quale ringrazio il collega, presidente Ostellari, che ha fatto un lavoro incredibile. Puniamo pesantemente chiunque discrimini in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, alla razza, alla religione e ad altre condizioni. Io voglio che, dopo il Covid-19, l'Italia sia un Paese bello, libero e tollerante. Rispetto chiama rispetto. *(Applausi)*. Colleghi, io vi chiedo di togliere dal banco, una volta per tutte, quello che divide. In un mese, sia il Senato che la Camera devono approvare una norma di civiltà che punisca pesantemente chi offende, aggredisce o discrimina un altro essere umano, perché in questo Paese nessuno è superiore a nessun altro. Andiamo, dunque, a votare questa legge. Se, invece, qualcuno, per tenere unito il proprio partito, che rischia di dividersi in 18 correnti, non vuole che *gay*, lesbiche e trans siano tutelati, lo dica ad alta voce in questa Aula. La Lega e il centrodestra vogliono risolvere i problemi. Chiudiamo qui la questione e approviamo tutti insieme la legge che questo Paese si merita. Vi ringrazio e aspetto e spero una risposta positiva.

che possano essere puniti coloro che discriminano, innanzitutto bisogna, non solo essere coerenti -ma la coerenza, si sa, non è di questo mondo - ma anche sapere quello che si dice e quello che si scrive.

appare assolutamente - questo leggo - decontestualizzato estendere tale previsione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, aggiungendoli all'elenco delle discriminazioni

possano essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione. Pertanto, le disposizioni di quella legge sacrosanta che prevede che debbano essere punite le discriminazioni per motivi razziali, etnici,

discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere. Ribadisco che l'identità di genere viene indicata con chiarezza in ben due sentenze della Corte costituzionale. sede, invece, si fanno dei film sull'interpretazione filosofica e antropologica dell'identità di genere, quando invece ci troviamo davanti a un fatto semplice: noi vogliamo una legge che aumenti i diritti,

esattamente il contrario, perché vuole minare proprio i fondamenti della legge. Dico anche un'altra cosa, sempre al senatore Renzi.

non si dovevano fare. Lo dico sempre a onor del vero, perché questo è. Allora oggi il nostro senso di responsabilità non è quello di fingere di fare una mediazione in di fingere di fare una mediazione in questa sede e modificare la legge. Adesso tutti credete al fatto che poi alla Camera in poco tempo si fa, quando gli articoli su cui si sono concentrate tutte le critiche erano frutto proprio di

della collaborazione delle famiglie. È già tutto scritto e specificato. Non usiamo quindi pretesti: andiamo avanti perché credo che possiamo fare un grande lavoro per le tante persone, uomini e donne, che in questo momento non hanno alcuna difesa. ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento,